in particolare, i senatori eletti in Veneto, signor Presidente, hanno letto stamattina che il governatore altoatesino, Luis Durnwalder, ha dichiarato tutto il suo favore e il positivo accoglimento da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo....

quella parte del comma 1 che, come prima abbiamo sottolineato all'Assemblea, pone in capo agli ispettori del lavoro la facoltà di sospendere l'attività produttiva nel caso di violazioni del lavoro straordinario. Segnalo davvero all'Assemblea, ancora una volta, la gravità di tale disposizione il fatto che si arrivi ad interrompere l'attività produttiva in presenza di una violazione rispetto alla quale, quantomeno, può ritenersi non proporzionata la sanzione. Aggiungo che, a differenza di analoghe disposizioni recentemente introdotte per quanto riguarda violazioni del rapporto di lavoro, in questo caso nemmeno si considera l'eccezione, altrove appunto considerata, relativa alle attività agricole e al loro ciclo ciclo biologico, che non può essere interrotto se non si vuole compromettere definitivamente la vita stessa dell'impresa. Io credo che questa disposizione sia davvero grave, prego il rappresentante del Governo di riconsiderare il suo parere negativo e chiedo a tutti i parlamentari, a tutti coloro che non sono viziati da una lettura ideologica del problema, di condividere questo emendamento e di rimuovere una odiosa disposizione le cui conseguenze potrebbero davvero essere gravi per molte imprese e per molti lavoratori che sarebbero i terzi incolpevoli in questo caso.

di una cosa di cui non si dovrebbe nemmeno parlare, nel senso che è ovvio, per chi lavora, che ci sono delle situazioni in cui, evidentemente, alcune cose sono semplicemente obbligatorie. È ovvio che, per esempio nel caso delle aziende agricole, ci sono le stagioni in cui si succedono avvenimenti naturali particolari che certo non possono essere gestiti in maniera programmata e distribuita durante tutto l'arco dell'anno lavorativo. Non si possono fare piani quinquennali dappertutto, contrariamente a quanto qualcuno nella maggioranza pensa ancora, per cui ci sono delle situazioni in cui, semplicemente, la giornata lavorativa non può essere di otto ore e la settimana lavorativa non può essere di cinque giorni. Devo dire che è imbarazzante essere in quest'Aula per dire cose talmente ovvie che se qualcuno fuori ci sentisse

ragioni, distanzia sempre di più dal Paese il mondo dei rappresentanti del popolo (teoricamente), il Palazzo, che dovrebbe fare cose di buonsenso e migliorare la vita dei cittadini mentre invece, alla fine, produce solo provvedimenti burocratici

stabilendo nella Costituzione che il matrimonio è l'unione fra più individui e non va bene quando invece permette di liberalizzare l'orario di lavoro. Non si può volere sempre tutto e il contrario di tutto.

legislativo n. 626 del 1994 e dell'inasprimento che viene portato, con l'articolo 2, alla disciplina già da tempo introdotta a seguito dei decreti

n. 626 avevano determinato negli anni passati, a stretto ridosso degli anni d'approvazione, quindi 1994, 1995 e 1996, una certa difficoltà per l'adeguamento da parte delle imprese agli stretti regimi di sicurezza che venivano a suo

alla necessità di introdurre dilazioni in ordine all'introduzione delle disposizioni concernenti questa tipologia.

quest'enorme attenzione, questa scarsa mancanza di prudenza nel prevedere pene e sanzioni abbia un effetto depressivo rispetto all'energia all'energia che in questo momento si sta sviluppando nel Paese, alla capacità di ripresa e ad un nuovo interesse per poter intraprendere e per poter produrre Credo sia un provvedimento molto squilibrato dal lato della sicurezza da garantire al lavoratore dipendente, mancando la necessità necessità che tutto questo sia contemperato con una certa prudenza per l'introduzione di norme che hanno un peso eccessivo nei confronti del datore di lavoro e dell'impresa.

Questa farraginosità e questa eccessiva attenzione agli organismi paritetici, la loro costituzione, la valutazione dell'applicazione delle vigenti norme rappresentano una complicazione enorme ed incredibile;

la sicurezza dei lavoratori se questi non hanno di che esserci: infatti, se non esiste la possibilità di lavoro e l'incoraggiamento ad intraprendere, non avremo dipendenti da difendere quanto alla sicurezza sul lavoro.

l'introduzione di una revisione dei temi della sicurezza di cui all'articolo 2 contengono tutti i motivi per dichiararci contrari all'approvazione dell'articolo 6.

è semplicemente partitico, e non ci si può che rallegrare di norme di questo genere, perché ogni volta che c'è un'elezione voi colleghi della sinistra scoprite che esiste il Nord, di cui non siete in grado di interpretare

bastasse che il presidente del Consiglio Prodi si facesse vedere a mangiare pane e salame su un battello sul Po e immediatamente le popolazioni del Nord sarebbero accorse plaudenti e avrebbero votato per l'Unione;

Ricordo che in Italia ci sono 8 milioni di partite IVA, la maggior parte delle quali sono al Nord: se è possibile, vi odieranno ancora di più per una norma di questa natura. Dovremmo essere contenti perché - come diceva il collega Galli - forse capiranno di che pasta siete fatti, forse capiranno che non riuscite ad interpretare lo spirito delle classi produttive del Paese.

Non bastava la Guardia di finanza, non bastava l'Ispettorato del lavoro, non bastavano i Vigili del fuoco, non bastavano le ASL: vi inventate un altro organismo - che peraltro esiste già ma se ne sta per il momento a casa propria - che ha poteri ispettivi e addirittura di denuncia; quindi se ne andranno in giro anche in questo caso e, visto che hanno questo nuovo potere, lo eserciteranno. Si andrà a vessare ancor più le piccole e medie aziende, gli artigiani, i commercianti e quant'altro. Mi domando come si possano scrivere simili norme.

perché va ad appesantire ancor più il corpo degli adempimenti e delle ispezioni che verranno effettuate a carico di chi cerca semplicemente di creare un po' di ricchezza per il Paese. Quanto

Quale è il significato di ciò? Quando si partecipa a una gara bisogna effettuare, ai sensi dell'articolo 7, lo splittaggio delle cifre che compongono il prezzo finale di offerta e il prezzo relativo alla sicurezza sul lavoro deve essere congruo.

caso in cui ci si aggiudichi la gara anche tenuto conto delle offerte anomale (perché sono molteplici i sistemi di aggiudicazione e non soltanto quello con l'esclusione delle offerte anomale), nel caso in cui cioè, indipendentemente dalle offerte anomale, ci aggiudichi la gara al massimo ribasso, l'articolo 7 non ha significato in quanto si può benissimo lasciare invariata la cifra relativa alla sicurezza sul lavoro e procedere a un ribasso ben superiore sulle

L'emendamento 8.201 ripropone il tema della proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni. Come abbiamo già visto in altre parti del provvedimento, il criterio della proporzionalità non è stato per nulla seguito, con la conseguenza di un'insufficiente effettività

nelle attività marginali, in tutto o in parte sommerse, per le quali l'inasprimento della sanzione risulta davvero inefficace,

la rubrica prevedendo l'omicidio doloso e le lesioni dolose e di conseguenza modificando gli articoli di riferimento del codice penale, in modo che le sanzioni disposte abbiano un'effettiva proporzionalità con il tipo di reato commesso, che non può non avere carattere doloso per essere sanzionato nei termini quiprevisti. È un tema che si è riproposto anche in precedenza: vogliamo sottolineare come la sanzione debba aggravarsi quando appunto si ravvisa tutta l'intenzionalità necessaria in colui che commette la violazione.

inasprire la sanzione pecuniaria di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, con la riscrittura dell'articolo 8 nella predisposizione proposta dalla Commissione la sanzione pecuniaria era stata portata a 400 quote. Oggi il Governo, in Aula propone di alzarla a 1.000 quote. Vorrei far osservare che si tratta di una filosofia che la maggioranza sta applicando non soltanto all'interno di questo provvedimento, ma anche dei precedenti, volta ad un eccessivo inasprimento nei confronti dell'imprenditore. Ricordiamo che

una previsione inerente al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che comporta addirittura la chiusura o il sequestro dell'azienda. E in base a quale previsione? In base all'articolo 589 del codice penale, che parla di omicidio colposo. Posso capire che, nel caso in cui vi sia un decesso, si possano applicare pene così terribili, ma l'articolo 590 parla di lesioni gravi; ciò significa che verifica un incidente, come ne accadono purtroppo ancora a migliaia nelle aziende italiane, il magistrato in caso di condanna può addirittura sequestrare l'azienda. Con quale modalità? Mettendo in luogo del datore di lavoro, dell'imprenditore o del dirigente un uomo di sua nomina. Siamo praticamente all'esproprio proletario da parte di Magistratura democratica. Questo è il quadro. Vedo che qualcuno sorride, ma c'è da piangere; c'è veramente da piangere. Stiamo portando avanti norme di questa natura che riguarderanno migliaia di aziende, perché purtroppo sono migliaia gli incidenti. Francamente non riesco a capire come possano essere state approvate in Commissione norme del genere. Il testo originario del Governo era tutto sommato equilibrato; mirava a costruire un testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ed era abbastanza condivisibile nei principi. Dalla Commissione è uscito un mostro che avrà conseguenze molto gravi sulla competitività delle nostre aziende. Diamo un altro colpo al sistema Italia con pene con pene veramente sproporzionate. Stiamo parlando di delitti colposi che sono evidentemente di ben altra natura rispetto a quelli dolosi. Questo è ciò che stiamo per votare. Vedo un'indifferenza totale dell'Aula perché,

per i colleghi dell'Unione i soldi e le finanze in Italia sono come la manna: scendono giù dal cielo, non nascono dal lavoro nelle fabbriche e nelle officine. Questo è il dato, però a voi non interessano per nulla questi discorsi: l'importante è scrivere norme vessatorie, l'importante è che ci sia qualcuno vessato, in modo da poter andare a casa tranquilli e dire: «Abbiamo fatto una bella norma che va a colpire i cattivi che fanno gli incidenti in fabbrica». Ricordatevi che la fabbrica a zero incidenti è quella chiusa; la fabbrica chiusa non è pericolosa, ricordatelo: fa zero incidenti, incidenti di nessuna natura.

dichiarare il voto contrario all'articolo 8 che per l'appunto, come era stato detto precedentemente, ha l'intento di aggiungere sanzioni accessorie per casi per cui già le norme attuali prevedono, com'è oltremodo giusto, la punizione dei colpevoli, oppure per comportamenti che in realtà non sono connessi a lesioni o

delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e non in conseguenza. Infatti, se in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche

dal relatore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 9.800 (testo 3), trasmesso all'Assemblea e relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

del credito d'imposta, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione di lavoratori a programmi e percorsi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un atto di regressione da parte dell'Assemblea in riferimento a quanto votato e deciso in Commissione. Commissione. Mi rendo conto che questo testo ha in qualche modo migliorato un precedente testo del Governo, però mi sembra che l'attesa dell'Aula fosse ben altra e non quella di compiere sforzi tali da ridurre il meno possibile le scelte già assunte in Commissione. Vedo che l'Aula del Senato ha preso una direzione molto negativa: si vive un clima completamente diverso da quello che c'è stato in Commissione. Invito pertanto il Governo a ritirare questo emendamento e a fare in modo che questa cifra vada a sostegno di ulteriori iniziative. C'è già un emendamento, votato dalla Commissione, che prevede 25 milioni di euro

Capisco anche che in proposito vi è un ordine del giorno del collega Barbato, ma non credo si possa andare avanti su temi come questi con ordini del giorno, nonostante il rispetto che merita l'iniziativa del collega Barbato. Il Governo si deve decidere: si sta parlando continuamente della necessità di intervenire su un punto così importante e puntualmente il Governo non lo fa. fa. Desidero denunciare tale atteggiamento e mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, che tanta sensibilità hanno mostrato, al presidente Treu e al relatore Roilo, che pure hanno mostrato grande sensibilità. Non riesco Non riesco a capire come il Governo possa procedere in un'operazione siffatta, dietro il titolo secondo il quale non ci sono fondi. Ma allora, se non ci sono fondi, pensiamo anche noi per il 3 per cento, per il 4 per cento a quel tesoretto di cui tanto si parla, ultimamente diventato il doppio o il triplo di quello che sembrava essere fino a qualche giorno fa. Come si può non rispondere ad esigenze così importanti e pregnanti, dicendo che non vi sono disponibilità? Stiamo parlando di pochissime e minime cifre. Allora, sollecito il Governo a ritirare questo emendamento

tre mesi che riempiamo i giornali, facciamo trasmissioni, si scomoda il Capo dello Stato per parlare di un problema che oggettivamente è serio. Parliamo di 1.500, 2.000 morti ogni anno, che in gran parte potrebbero essere evitati semplicemente con maggiore prevenzione, maggiore controllo o maggiore attenzione da parte delle stesse persone che lavorano. Poi facciamo tutta una serie di sproloqui in Aula sull'importanza della cultura, dell'informazione. Facciamo un intervento giusto per dare una nuova possibilità alle aziende che. comunque, devono investire dei soldi: se si svolge un corso di formazione durante l'orario di lavoro, credo che anche quelli che pensano che i soldi crescono sugli alberi capiscano che, se una persona per cinque ore segue un corso

ma tali questioni semplicemente non dovrebbero essere nemmeno quantificate, intanto perché la frazione di eventuale perdita fiscale è talmente bassa rispetto rispetto alle anomalie della contabilità dello Stato italiano che comunque nessuno sarebbe mai in grado di rilevarla, ma quand'anche fosse significativa non si può quantificare

onere annuo, con una maxicopertura, ma con dei problemi riguardo alla legge di contabilità. La proposta è stata variata, come lei vede, prevedendo una necessità di risorse per due anni e con una copertura diversa rispetto alla maxicopertura tipica, prelevando dal gettito delle accise sui tabacchi. Qual è il problema che rileviamo politicamente? In primo luogo, indipendentemente dalla difficoltà di copertura, la riduzione della cifra non tiene conto di un argomento su cui tutti ci siamo trovati d'accordo. Non ci si è trovati d'accordo sull'eccessiva garanzia, eccessiva non perché non meritevole o perché problema di fattore igienico nei confronti dei lavoratori, ma eccessiva rispetto ai tempi e alle modalità di introduzione come garanzia nei confronti del lavoratore. Non ci siamo trovati d'accordo sugli obblighi e le previsioni di sanzioni e di una disciplina sanzionatoria nei confronti dell'imprenditore, in quanto eccessiva o troppo veloce nel tempo. Una questione invece, su cui tutti ci siamo trovati d'accordo è la necessità della formazione, vuoi per i lavoratori, vuoi per i datori di lavoro.

si era trovata una soluzione senza necessità di copertura con la previsione di destinare il 5 per cento dell'insegnamento a materie tecniche o tecnico-giuridiche, ad esempio, con la famosa materia di applicazioni tecniche o con le materie giuridiche in istituti ove è previsto l'insegnamento del diritto, come possono essere quelli che avviano alla collaborazione societaria, come quelli per ragionieri o anche la scuola per geometri. Tutto ciò, invece, con una motivazione che non abbiano ben capito e con una difficoltà notevole è stato negato, ma per fortuna, comunque, approvato lo stesso dall'Aula da una parte della maggioranza. Ora ci ritroviamo con una diminuzione della copertura da 25 a 20 milioni di euro, con una diminuzione necessaria del periodo, per via dei problemi relativi ai sistemi di copertura e alla legge di contabilità, e con un periodo che non arriva neanche ai tre anni - circostanza che era possibile - e che si ferma al solo biennio. Capisco che la difficoltà possa essere costituita dal fatto che, Presidente, l'emendamento prevede che le spese sostenute siano per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Non ho letto esattamente, perché tra la parola "percorsi" e la parola "di", che precede "carattere formativo" c'è in realtà la parola "certificati". La verità sostanziale è che probabilmente il Governo non ha molta fiducia di come questi percorsi formativi possano essere certificati, di cosa significhi certificati, di come la mancanza di certificazione non efficiente comporti degli spazi di cattiva utilizzazione delle risorse per percorsi di formazione che invece di essere effettivi sono un sistema per parcheggiare o distribuire prebende e per dare la parvenza di una formazione, come quella a veline o a parrucchieri, di cui tanto si eccede in Regioni e Comuni di tutta Italia, in particolare - ahimè - del Meridione.

in specie da autorevoli Capogruppo della maggioranza. Poi invece su una proposta del genere, che è abbastanza prudente e limitata un percorso che dovrebbe trovarci tutti consenzienti, abbiamo questa rigidità del Governo che ci lascia ben capire quale deve essere nel prosieguo il nostro atteggiamento.

un roboante soffermarsi in sede legislativa - e non solo in sede legislativa, ma in tutte le sedi istituzionali - sulla questione vera e drammatica degli infortuni e delle morti bianche.

Cioè, con le sanzioni interdittive, si chiudono le aziende, si sequestrano i macchinari, si arrestano gli imprenditori, si multano per 500 euro gli operai che non ostentano il cartellino, però mentre l'operaio deve pagare 500 euro se non ostenta il cartellino, allo stesso tempo lo Stato bada a risparmiare 5 milioni di euro nelle misure di prevenzione. Penso che in tale dato ci sia tutta l'ipocrisia non solo di questa maggioranza, non solo di questo Governo, ma anche dei lavori di quest'Aula,

e futuri, è l'elemento costitutivo delle moderne politiche del lavoro e delle moderne politiche ambientali. Ecco, Presidente, perché dissento dal mio Gruppo: perché il mio Gruppo non ha centrato la questione politica dell'opposizione su questo emendamento.

alla conoscenza delle regole preposte a garanzia dalla propria sicurezza». Questo ordine del giorno, dunque: «impegna il Governo ad incrementare le risorse per garantire maggiori investimenti sulla sicurezza sul lavoro e, in particolare,

nuova formulazione, introdotta dall'emendamento del senatore Tofani, restano l'obbligo e la possibilità di effettuare i controlli sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro anche alle imprese che hanno aderito a questa regolarizzazione del lavoro sommerso prevista dal comma 1192 della finanziaria.

che hanno aderito a questa regolarizzazione, a questa emersione del lavoro sommerso, sono esentate per un anno dai controlli, dalle ispezioni e dalle verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza, comprese quelle concernenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Allora è positivo che vi sia questo articolo, ma è estremamente negativo che a tutt'oggi sia in vigore una norma (ed è in vigore fin dall'inizio di quest'anno), introdotta dalla finanziaria di questo Governo, che esenta certe aziende che hanno fatto una regolarizzazione di carattere amministrativo, per per regolarizzare il lavoro nero e non per regolarizzare il lavoro in condizioni tali da mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. Credo che questo andrebbe sottolineato e andrebbe ricordato che a tutt'oggi, e finché questo o altri provvedimenti non verranno introdotti per modificarlo, il Governo e la maggioranza hanno messo in vigore e lasciano che sia in vigore una norma che esenta alcune aziende dai controlli sulla salute e sulla sicurezza del lavoro. Credo che questo, da parte di una maggioranza che ebbe molto da ridire sui condoni, unicamente di carattere fiscale, proposti dal Governo precedente, proposti e votati dalla maggioranza precedente e che avevano unicamente conseguenze di carattere fiscale (e peraltro hanno ottenuto il risultato di far pagare le tasse a chi non le pagava), da coloro che hanno criticato quei condoni, che parlavano, alla fin fine, di vil denaro (al quale dobbiamo rispetto, ma non certo pari a quello che dobbiamo alla salute dei lavoratori), hanno introdotto il condono delle violazioni a danno della salute e della sicurezza dei lavoratori.

al fatto che dice in quest'Aula che non ha fatto condoni e non farà più condoni, non vorrei correre il rischio che l'accalorato intervento del senatore Malan convinca molti colleghi della maggioranza a votare

correzioni e condoni, come nella fattispecie. Fra le altre cose, è pur vero che questo condono è assolutamente scandaloso, quindi voterò in modo tale da rendere evidente che il Governo

(testo 2) sostituisca con l'utilizzo di un accantonamento di fondo speciale del Ministero dell'economia un prelievo fiscale aggiuntivo che non avremmo potuto condividere ancorché riferito ancora una volta all'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico. Credo si debba rinunciare sempre all'inasprimento fiscale perché i livelli di pressione fiscale sono comunque pervenuti ad un grado tale da non consentire ulteriori aggravi, anche quando le ragioni possono essere nobili come sono quelle relative alle assunzioni di ispettori del lavoro a valere su un concorso che il Governo del quale ho avuto l'onore di fare parte ha promosso ed espletato. Rimane la necessità di completare l'assunzione di tutti gli idonei del concorso, ma - come ho detto - questo in ogni caso non può che essere considerato un passo in avanti: dai Gruppi di opposizione in Commissione e pertanto non può non essere sottolineato il fatto positivo di un rafforzamento del numero degli ispettori del lavoro.

significa, di fatto, non assumere 600 idonei, ma assumerne 300, vale a dire tagliare la metà degli idonei.

cui l'Assemblea non sta migliorando il provvedimento, ma lo sta fortemente minando, addirittura riducendone l'efficacia. Pertanto, chiedo che venga espresso un voto contrario e e non comprendo chi è d'accordo con un emendamento del Governo che di fatto riduce la possibilità di assumere gli ispettori per i controlli, per la prevenzione e per la repressione di casi che dovessero essere *contra legem* sui posti di lavoro, per dare una risposta alla sicurezza sul lavoro. Mi auguro, colleghi senatori, che nella severità dei vostri sentimenti e nella onestà intellettuale che vi contraddistingue, che comunque ci deve contraddistinguere, possiate respingere questo emendamento del Governo, che tra l'altro è una provocazione.

venire in Commissione e in Aula a spiegarci come sono tutti brutti e cattivi quelli che fanno impresa e come fortunatamente ci siete voi della maggioranza a difendere i lavoratori, poi di fatto, quando si arriva al momento della decisione, al dunque, tirate via quattro soldi che servono per la prevenzione, dite che servono più controlli e non fate passare l'assunzione dei nuovi ispettori. Quindi, nella vostra logica effettivamente si fa fatica

che non si tratta di continuare ad assumere persone. Con la legge finanziaria 2007 avete regolarizzato 500.000 dipendenti pubblici precari, cioè a tempo determinato, facendoli diventare a tempo indeterminato; questo porta, tra dipendenti pubblici a tempo indeterminato (che ormai sono la stragrande maggioranza), quelli rimasti a tempo determinato e tutti quelli che non vengono contati come dipendenti pubblici ma che di fatto lo sono, a quasi 5 milioni di persone,

per qualunque tipo di lavoro sono state fatte con concorsi dove partecipano molte persone, quindi, per esempio, la stragrande maggioranza degli assunti, indipendentemente dal lavoro che andranno a svolgere effettivamente, sono comunque laureati praticamente in tutte le materie esistenti nei corsi di laurea universitari del nostro Paese. Quindi, la pubblica amministrazione deve mettersi a guardare al proprio interno e tirar fuori di lì le risorse che servono per affrontare i problemi che diventano più importanti nel Paese. Che si tiri via qualcuno dalle ex Partecipazioni statali, che si tiri via qualcuno dalla Camera e dal Senato, che negli ultimi vent'anni hanno aumentato del 50 per cento i loro dipendenti,

i soldi non crescono sugli alberi! L'altro giorno avete aumentato gli indici degli studi di settore per far pagare più tasse a quelli che già le pagano e poi sprecate i soldi in questa maniera: non è una cosa accettabile! Se vogliamo essere un Paese moderno, non lo si fa con i *tour* sul Po o con quello che ha detto Veltroni mezz'ora fa a Torino, ma con i fatti. I Paesi seri equivalenti al nostro, quando hanno troppi statali, li licenziano; quando hanno un'esigenza li riqualificano, e nessuno si scandalizza per questo. Se assumiamo una persona è a vita; se è assunto a fare un lavoro che poi, dopo due anni, non c'è più, per i successivi quarant'anni continua a svolgere quel lavoro e a prendere lo stipendio. Credo non ci sia nulla di scandaloso a dire ad un dipendente statale, che magari sarebbe anche più contento di svolgere una mansione utile, che il suo lavoro non serve più, che si fa un anno di riqualificazione e lo si mette a fare qualcos'altro: sarebbe più serio nei confronti del dipendente pubblico pubblico ed enormemente più serio nei confronti del Paese. Magari non dovremmo assumere i 300 ispettori che non so alla fine se assumerete o no, magari ne troveremmo 2.000, che sono molti di più e che farebbero altrettanto bene, sei volte di più, il lavoro di ispezione se è diventato più importante rispetto ad altri.

un appello anche alla coerenza dei colleghi della cosiddetta sinistra radicale. Loro sostanzialmente hanno votato a favore di un emendamento che colpiva le politiche di prevenzione. Ora siamo qui a vedere se voteranno a favore di un emendamento che colpisce le politiche di controllo. Prevenzione e controllo sono infatti di qualsiasi attività seria diretta a limitare gli infortuni sul lavoro e le cosiddette morti bianche. Staremo a vedere ora se la sinistra radicale sarà coerente con quanto sostiene fuori dal Parlamento.

l'aumento dell'età pensionabile a 62 anni per le lavoratrici, tra il silenzio e la complicità del sistema mediatico e anche della sinistra radicale; non mi risulta che qualcuno di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani di Diliberto si sia opposto a quanto andavano ventilando i giornali circa l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 62 anni; non mi risulta che si sia levata una voce da questo Parlamento. Così come non mi risulta che oggi in questo Parlamento ci sia una voce da parte della sinistra radicale,

di grida manzoniane e di proclami, di temi suggestivi da agitare di fronte all'opinione pubblica, allora si è quanto mai radicali, ma poi nel concreto, qui in Aula e non solo, ma anche a Palazzo Chigi, allora non si è nemmeno riformisti, ma soltanto

compiuta nell'arco di sei mesi la più grande operazione di investimento per una figura che è necessaria in particolare per ciò che riguarda

perché, da un lato, per quanto riguarda gli ispettori del lavoro prevede l'assunzione degli idonei e, dall'altro, al Ministero delle finanze, nega la medesima scelta. È stato deciso, infatti, di procedere ad un nuovo concorso frustrando le aspettative di migliaia di giovani che avevano partecipato a selezioni difficili, garantendo così la copertura di posti importanti nell'Amministrazione finanziaria per la lotta all'evasione a supporto delle politiche tributarie del Governo. Il Governo ha preferito invece

in merito alla richiesta del Comune di Cortina d'Ampezzo di aderire alla Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige. Tutto ciò avviene dopo che altri Comuni situati nei confini della Regione Veneto hanno segnalato, addirittura ottenendo durante il *referendum* consultivo delle popolazioni ampi consensi, il tema

Adige. Al riguardo spiace molto dover registrare che le dichiarazioni del presidente Durnwalder non siano per nulla rispettose, invece, di una questione che sta diventando sempre più spinosa, ma sulla quale la Regione Veneto non potrà continuare a restare passiva. Dopo Lamon e Sopramonte, dopo i sette Comuni dell'Altopiano di Asiago e Portogruaro, per noi oggi la questione di Cortina è quanto mai importante. Le chiederei quindi di poter far intervenire il Governo in quest'Aula

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, finalmente, per merito del Presidente della Repubblica, la mancata sicurezza sul lavoro è entrata nell'agenda politica del nostro Governo e del nostro Parlamento. Le premesse politiche contenute nella legge finanziaria per il 2007, che con il comma 1198 garantisce la sospensione di un anno dei controlli sulla tutela della salute e della sicurezza nelle aziende che manifestano l'intenzione di regolarizzare lavoratori prima in nero, non lasciano ben sperare; così come la scelta di sviluppare le assunzioni degli ispettori del lavoro con funzioni amministrative, non dando invece la necessaria priorità a quella dei tecnici del lavoro, la cui mancanza di controllo degli impianti produttivi e dei luoghi di lavoro è al momento l'anello più debole di tutta la catena. Tuttavia, la vicenda di Matteo Valenti, il ragazzo di 23 anni morto sul lavoro a Viareggio, è lì a gridare che non è solo la politica a segnare un fortissimo ritardo di cultura e di civiltà, ma che l'insieme della nostra organizzazione sociale ha lasciato passare una sorta di irresponsabile fatalismo. La persona responsabile di quell'omicidio sul lavoro, mentre ha riconosciuto la sua colpa patteggiando una condanna a 20 mesi (con l'indulto, ovviamente, lo hanno subito liberato), non solo non ha sentito il dovere di dimettersi da presidente provinciale dei commercianti, ma all'indomani del patteggiamento ha addirittura utilizzato tale carica rappresentativa per far uscire un comunicato ufficiale della sua associazione presentandosi come vittima di una immotivata persecuzione. Era perseguitato con tanto accanimento che, mentre era imputato di omicidio, la Cassa di risparmio di Lucca, Pisa e Livorno ha pensato bene di fare cosa buona e giusta chiamandolo a far parte del proprio consiglio d'amministrazione. Alla sicurezza sul lavoro occorre affiancare la sicurezza del lavoro, nonché il riconoscimento del ruolo essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori nella vita economica, sociale e culturale del Paese. Gli impegni morali in questa materia, per il rispetto che a quei morti è dovuto, debbono tradursi in atti e scelte precise. Le mie proposte sono un concreto aumento delle risorse che devono andare al potenziamento degli ispettorati del lavoro una revisione dell'attuale tendenza dell'INAIL a ridurre le proprie tabelle per l'invalidità e per la morte sul lavoro. Le multe, inoltre, che le ASL applicano per il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni vadano in gran parte utilizzate per aumentare l'esiguo numero di addetti a tale servizio. Stato, Regioni ed enti locali individuino forme premiali per quelle imprese che, andando oltre le attuali norme di legge, adottino ulteriori innovazioni di processi e di prodotto in grado di elevare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che andrebbero però eletti dai lavoratori a cui debbono rispondere e non nominati dai dirigenti sindacali. Il mio voto non mancherà, pur mantenendo una posizione fortemente critica su ciò che è stato fatto fino ad oggi e sperando che l'impegno del Governo e dell'Unione abbia una decisa impennata.

il proficuo confronto tra operatori, studiosi ed amministratori ha permesso di individuare le priorità di un programma coerente di riforma in materia di sicurezza sul lavoro. Dunque, vi è ora l'impellenza di un riassetto che sintetizzi la normativa dagli anni Cinquanta ad oggi, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e dell'equilibrio tra Stato e Regioni. Grazie a questa delega l'Esecutivo potrà approvare un testo unico la cui stesura mi auguro sia completa disciplina a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il dibattito politico, preludio della formulazione legislativa anche innovativa, deve necessariamente tener conto sia dei diritti sia dei canoni di sicurezza di ambedue le parti del rapporto di lavoro. Si tratta di un passaggio di grande valore a fronte delle evidenziate carenze dell'attuale panorama normativo in materia di sicurezza e delle cifre allarmanti di morti e infortuni

trasposta nelle linee guida oggi al vaglio. Il documento ha, infatti, ampi margini, entro cui spaziare, dettati da criteri che, benché generici, rappresentano la giusta guida per l'Esecutivo. Mi voglio brevemente riferire ad alcuni validi principi e criteri direttivi contenuti nella delega, cioè ai presupposti da fornire alle aziende circa la relazione e la diffusione di codici di condotta, primo passo per garantire e innalzare i livelli di tutela. E, proprio con riferimento alle misure a sostegno delle imprese e finalizzate alla formazione dei dipendenti ed alla conoscenza delle regole preposte a garanzia della loro sicurezza, voglio sottolineare l'accoglimento, da parte del Governo, dell'impegno contenuto in un ordine del giorno a mia firma, che auspica il rafforzamento della previsione contenuta nell'articolo 9, così come modificato dall'Assemblea. La disposizione in questione prevede la concessione di un credito d'imposta ai datori di lavoro nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro. Mi auguro che il responsabile impegno del Governo ad aumentare lo stanziamento previsto possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Tra i principi positivi, contenuti nella legge delega che ci accingiamo ad approvare, vorrei fare poi menzione alla razionalizzazione del sistema pubblico di controllo ed alla riformulazione dell'apparato sanzionatorio vigente, affinché si elevino le competenze e si ponga un forte deterrente alla violazione delle regole di sicurezza. Non a caso la 2a Commissione, che propone l'assorbimento dei disegni di legge

totale sproporzione tra le sanzioni - anche quelle di tipo esclusivamente amministrativo - e la gigantesca normativa cui sono poste a tutela, incoraggiando vivamente di adottate soluzioni deterrenti più idonee. Occorre perciò una netta valutazione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, ma anche sui potenziali pericoli per la popolazione. Occorre introdurre misure tutelari più energiche per specifiche tipologie di lavoro, in base alla particolare nocività di taluni ambienti. Occorre riservare una particolare attenzione al lavoro precario ed al *mobbing*. Occorre, infine, ridefinire i criteri qualitativi e quantitativi della formazione degli organi di vigilanza e della sorveglianza sanitaria. In conclusione, queste sono le più più che valide ragioni del nostro voto positivo. *(Il

economiche per realizzarle. Spero che questo provvedimento apra anche la possibilità di riprendere la discussione su un altro disegno di legge, di cui il senatore Casson è primo firmatario,

Tutte le indicazioni ci dicono che soltanto rafforzando il loro potere e la loro capacità di intervento, sarà possibile ridurre drasticamente gli incidenti sui luoghi di lavoro. Mi dispiace che l'Assemblea abbia respinto alcuni emendamenti che abbiamo presentato in tal senso e mi dispiace anche che altri emendamenti, soprattutto del Gruppo Verdi-Comunisti italiani, non siano stati approvati. Devo dire, peraltro, che gli esponenti di questo Gruppo non li hanno difesi, come credo sarebbe stato giusto adeguatamente in questa sede fare ma che io, però, ho votato.

possano restare anche eventualmente lettera morta, se non si accompagnano a qualcosa di strettamente correlato. Mi riferisco, in particolare, ad un intervento sulla precarietà, sulle leggi che hanno creato e determinato la precarietà. In Aula ed in Commissione moltissimi hanno sottolineato che l'elemento della sicurezza del lavoro è fortemente collegato alla stabilità, alla sicurezza in senso più generale del posto e che la precarietà è una delle fonti principali degli incidenti. Su questo, ad un anno e più di distanza dall'insediamento di questo Parlamento, nonostante le promesse e gli impegni fatti, ancora non si è fatto nulla praticamente o molto poco; cose molto limitate seppur importanti in finanziaria, ma non un provvedimento organico legislativo. Da questo punto di vista non mi rassicurano affatto le indiscrezioni le indiscrezioni che leggo sui giornali rispetto alle proposte del Ministro del lavoro sulle leggi della precarietà, che mi paiono ultraridotte, limitatissime e che non interverrebbero, se restassero tali, sulla questione di fondo, cioè su un superamento drastico della legge n. 30 e di tutte le leggi che hanno determinato la precarietà. Resterà lettera morta anche questa legge se non operiamo sul terreno di un intervento fortissimo in questa direzione. Infine, penso anche, penso anche, come avevo già sottolineato nell'intervento in corso di discussione generale, che deve mutare anche il clima nel Paese rispetto alle organizzazioni sindacali, rispetto al mondo del lavoro. Se la centralità è soltanto l'impresa, il lavorare di più, il ridurre i costi del lavoro, ridurre i tempi, aumentare gli orari di lavoro - perché questo è quanto avvenuto concretamente nel corso degli ultimi anni - ebbene, gli incidenti non solo non diminuiranno, ma continueranno ad aumentare. Se non cambia la percezione complessiva nel Paese e tornano ad essere al centro i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, veramente il diritto al lavoro ma anche alla sicurezza del lavoro - e questo passa attraverso un riconoscimento pieno di nuovo di un protagonismo del mondo sindacale e del mondo del lavoro - sarà molto difficile affrontare alla radice le cause che determinano le morti sul lavoro e che questa legge positiva che oggi votiamo possa realizzarsi fino in fondo.

La Lega Nord voterà contro questo provvedimento, come risulta evidente da tutti gli interventi che abbiamo fatto durante la discussione di queste giornate, non perché non non perché non ritenga esserci un problema nel nostro Paese riguardante la sicurezza sul lavoro, come purtroppo la statistica impietosa, numerica, quotidianamente ci ricorda, ma proprio perché questo provvedimento, che affronta un argomento estremamente importante, è partito nella prima stesura in maniera condivisibile: era un documento semplice, snello, che indicava solo princìpi generali, tra i quali soprattutto quello di armonizzare la legislazione e di ridurre gli eccessi burocratici, cioè di andare alla sostanza del problema e di diffondere, soprattutto, la prevenzione. modalità assolutamente condivisibile, che ci avrebbe visti favorevoli se durante il passaggio in Commissione, e poi anche in Aula, con peggioramenti in corso d'opera, non fosse stata completamente stravolta. Difatti, il testo che ne esce ha poco a che fare con l'intenzione originaria. È un testo che, di fatto, si è trasformato esclusivamente in un ulteriore appesantimento burocratico-legislativo

non accettabile le pene pecuniarie, senza peraltro affrontare il cuore del problema, che ovviamente non si può affrontare in maniera puramente legislativa e burocratica. Infatti, come detto e ampiamente spiegato da tutti i colleghi, in Italia il problema delle morti bianche non è legato a una mancanza di legislazione, che anzi nel nostro Paese è sicuramente tra le più severe del mondo occidentale. Fra parentesi, il mondo occidentale è l'unica parte del pianeta che si occupa di tale questione, perché, lasciamo perdere Paesi sottosviluppati a livello tale per cui di questi argomenti probabilmente neanche si può parlare, ma anche in Paesi che in realtà sono in grande

gli incidenti gravi, a livello statistico, non accadono più in misura rilevante nelle grandi aziende organizzate. Aggiungo di più, non accadono quasi più neanche nelle piccole, medie o piccolissime aziende,

dove i controlli non ci sono, dove magari lavorano persone non regolarmente assunte, dove magari i prezzi sono particolarmente tirati e le persone sono portate a lavorare in un certo modo, anche qui non per ragioni particolarmente difficili da interpretare.

anche di questo si dovrebbe parlare con altrettanta serietà. Però, effettivamente, per una ragione statistica, da anni ormai, gli incidenti sulla via del lavoro sono considerati infortuni e quindi, statisticamente, si ha questo risultato. Il resto avviene soprattutto nei cantieri per caduta dei ponteggi. Si cade dai ponteggi perché o manca la ringhiera, semplicemente, o perché non si usa la cinta di salvataggio con un collegamento ad un punto fisso sicuro. Queste cose non richiedono tutti gli interventi scritti in questo provvedimento, non richiedono di mettere in galera l'imprenditore che fa fare due ore in più di straordinario ad un tornitore che lavora su una macchina a controllo numerico che va da sola e dove il pericolo è pari a zero. Si risolve semplicemente amplificando, incrementando in maniera esponenziale i controlli dove avvengono gli incidenti. Se noi potessimo tenere sotto controllo i cantieri edili dove non vengono rispettate queste norme basilari di sicurezza, subito dimezzeremmo le morti bianche.

dove invece gli incidenti capitano. A questo proposito, il fatto di avere ridotto di cinque milioni, una cifra ridicola, su 25, che è altrettanto ridicola, la spesa per la prevenzione e avere ridotto di metà le assunzioni degli ispettori, per quanto riguarda il discorso che ho fatto prima,

Signor Presidente, per prima cosa vorrei evidenziare che noi abbiamo lavorato duramente in Commissione, ed è stato un lavoro molto proficuo, costruttivo, che il contributo dell'opposizione, del Governo e naturalmente della maggioranza. Un lavoro che, purtroppo, non si è rispecchiato in quest'Aula in cui ha prevalso la posizione politica, lo scontro politico, che su una materia così importante e che tutti condividono non era decisamente appropriato. Stiamo approvando un importante disegno di legge che delega al Governo il riordino della materia della salute e sicurezza sul lavoro. È un provvedimento importante perché mira a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, quelli autonomi e quelli dipendenti, prevenendo gli infortuni, puntando sull'educazione e su misure di precauzione per ridurre gli incidenti e le morti bianche purtroppo troppo frequenti anche nel nostro Paese. Noi, in Commissione, come dicevo, abbiamo dato un contributo forte, l'ha dato anche l'opposizione e c'erano tanti emendamenti del Gruppo Per le Autonomie che coincidevano con

senza ridurre la protezione né la sicurezza per i lavoratori. Questo è anche l'appello che faccio al Governo qui presente perché ne tenga conto. Abbiamo anche tenuto conto delle differenti situazioni, gli artigiani avevano proposto di togliere gli autonomi da questa legge, giustamente si è detto che anche all'autonomo serve una certa protezione, era però giusto differenziare tra situazioni di micro-economia e di micro-aziende, in cui l'artigiano lavora da solo, magari con sua moglie e i suoi figli, e un grande cantiere - com'è stato rilevato poc'anzi dal senatore che ha naturalmente più pericoli intrinseci all'operato. Abbiamo previsto

di aver proposto una mozione che era espressione dell'anima di quanto è successo in Commissione stessa, per aumentare i mezzi di 20 milioni per incentivi alle aziende, percorsi formativi, forme di credito d'imposta. Ricordo un ulteriore emendamento proposto dal mio Gruppo che ha potenziato il ruolo del medico competente, oltre a quello del rappresentante dei lavoratori. È previsto che nella commissione di prevenzione e monitoraggio sui luoghi di lavoro Grazie Abbiamo introdotto un nuovo concetto, anch'esso con emendamento del Gruppo per le autonomie: il riconoscimento giuridico degli accordi aziendali e dei codici di condotta etici, abbiamo lottato per questa introduzione, perché abbiamo detto che non era necessario fissare tutto nei decreti legislativi che dovranno seguire, è stato poi accolto poi accolto anche questo nostro emendamento. Siamo pertanto soddisfatti che il Senato rafforzi la prevenzione per la sicurezza, auspicando di diminuire con ciò gli infortuni e le tragedie sul posto di lavoro. Siamo anche soddisfatti che in sede di Commissione sia stato possibile coniugare, con questo principio, l'obiettivo di semplificare la materia e di tenere conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e di non appesantire troppo gli oneri burocratici. Ringrazio in questo senso il presidente Treu, che ha con grande pazienza e professionalità condotto i lavori, il relatore Roilo, i rappresentanti del Governo Patta e Montagnino. Ho già detto che sono contento che siano stati aumentati anche i mezzi, ho già citato quelli in forma di credito d'imposta per le aziende e ci sono altri 20 milioni in più per le assunzioni degli ispettori che avevano già vinto il concorso e pertanto anche qui c'è un aumento e non una diminuzione. Abbiamo apprezzato l'ordine del giorno che sollecita il Governo, mi appello al Governo nell'attuazione della delega di cercare di essere semplice, di non appesantire troppo per le piccole e medie imprese gli oneri, naturalmente sempre con l'obiettivo da una

onorevoli colleghi, di fronte all'aumento dei decessi legati agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali, l'Organizzazione mondiale della sanità e l'*International Labour Office* il 28 aprile hanno dedicato una giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro cercando di sottolineare la necessità di creare una cultura della prevenzione a livello globale. Secondo i dati forniti, il numero delle vittime causate da incidenti e malattie legate al lavoro supera i 2 milioni di unità ed è in crescita, in particolare a causa del processo di industrializzazione di molti Paesi in via di sviluppo. Inoltre, il rischio di malattie legate al lavoro è diventato sempre più grave: 1.700.000 decessi risultano essere causati ogni anno da malattie professionali. L'obiettivo di migliorare la salute dei lavoratori ha condotto l'Organizzazione mondiale della sanità a collaborare più strettamente sulla sicurezza occupazionale. L'Organizzazione mondiale della sanità sta aiutando le diverse Nazioni a mettere a punto strategie di prevenzione e ha istituito un *network* che raggruppa 70 centri collaborativi in tutto il mondo. Naturalmente questa premessa serve per comprendere in quale ambito culturale-politico e giuridico-amministrativo stiamo operando e - debbo dire - anche con un po' di ritardo. «A dispetto di significativi miglioramenti nella salute e nella sicurezza in molte parti del mondo, negli ultimi decenni l'obiettivo globale di garantire la salute e la sicurezza ai lavoratori è ancora lontano dall'essere stato raggiunto». Così sottolinea la direzione generale del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e l'ambiente sempre della stessa Organizzazione. Più in generale, è anche utile ricordare che nei prossimi 15 anni ci sarà un aumento sia del numero dei giovani che di quello degli anziani che entreranno nella forza lavoro e si sottolinea che si tratta proprio delle categorie che tendono ad avere i più alti tassi di incidenti sul lavoro. Ed è per tali motivi che si chiede la creazione di programmi di educazione e protezione specificatamente destinati a questi due gruppi. Dai dati diffusi dall'EURISPES, patrocinata dalla Camera dei deputati, le cifre sugli infortuni e sulla mortalità nel mondo del lavoro in Italia sono fortemente drammatiche e mettono chiaramente in risalto l'inefficacia dei provvedimenti legislativi a tutela dei lavoratori messi sinora in campo. Per rimarcare la triste portata del fenomeno delle morti bianche ha quindi fornito delle cifre allarmanti: dall'aprile 2003 (anno di inizio della seconda guerra del Golfo) all'aprile 2007 i militari della coalizione che hanno perso la vita durante le operazioni belliche sono stati 3.520; i morti sul lavoro in Italia dal 2003 all'ottobre 2006 sono stati 5.252. Quindi, dalla serie storica 2000-2006 risulta che ogni anno in Italia muoiono in media 1.376 persone per infortuni sul lavoro; poco meno del 70 per cento dei lavoratori (circa 850) perdono la vita per cadute dall'alto di impalcature nell'edilizia o per ribaltamento del trattore in agricoltura o ancora in un incidente stradale nel trasporto merci per le eccessive ore trascorse alla guida. colpiti da infortuni mortali si aggira sui 37 anni per cui, dato che l'aspettativa di vita alla nascita è in media di circa 79 anni, ogni incidente comporta una perdita di vita pari a 42 anni.

visibili. Per tali motivi, condividiamo l'urgenza che muove questo specifico provvedimento, ma per gli stessi motivi riteniamo assolutamente necessario porre in essere, almeno questa volta con l'appoggio sia della maggioranza che dell'opposizione, un provvedimento realmente incisivo e realmente definitivo.

di mettere in campo norme bilanciate. Tutto questo non ci induce a credere che esso sia realmente capace di raggiungere il fine proposto. Sicuramente non sufficienti sono le misure relative ai controlli sulla corretta applicazione della normativa stessa, che è il problema fondamentale della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non condividiamo, inoltre, lo strumento della delega. Sulla questione c'è ampia convergenza, una convergenza che avrebbe potuto portare alla creazione di un testo condiviso veramente, contenente provvedimenti immediatamente precettivi ed emanati direttamente dal Parlamento, giusta sede di discussione e di dibattito. Quello di cui abbiamo necessità è un provvedimento complessivo, incisivo, che rimetta ordine in modo definitivo alla normativa vigente, una normativa dalle molteplici sfaccettature e che tocca ambiti civili, sociali, economici. Non riteniamo, inoltre,

In primo luogo, con questa legge credo si possa anche intravedere, per così dire, un giro di boa rispetto ad una inversione di tendenza che dovrà poi essere completata da altri interventi, orientamenti politici, patti sociali tra le organizzazioni sociali che rimetta al centro la questione della dignità e del valore del lavoro.

apprezzo - e credo dobbiamo farlo tutti - gli avanzamenti che sono stati fatti anche rispetto al provvedimento originale, tant'è che si è partiti da un articolo unico e si è arrivati ad 11, ma soprattutto

alla tragicità della situazione che ci troviamo ad affrontare. Non possiamo nasconderci dietro al fatto che siamo forse superiori alla media a livello europeo e che quindi in altri Paesi si muore di più.

per la tutela. Voglio ricordare l'obbligatorietà del coordinamento regionale tra tutte le strutture e gli enti preposti alla vigilanza o alla tutela, che porteranno senza dubbio risultati positivi; il rafforzamento dei poteri e dei diritti dei responsabili della sicurezza, oltre agli interventi maggiori sulla formazione, sia quelli aziendali ma soprattutto quelli territoriali e soprattutto quelli di sito, perché i dati indicano che laddove lavorano i rappresentanti sindacali per la sicurezza e sono in grado di intervenire, l'incidenza degli infortuni è molto più bassa.

le commissioni tra azienda e organizzazioni sindacali, e quindi questo sarà senza dubbio un passo importante. Così pure è importante intervenire e aumentare gli strumenti di prevenzione:

può illudere che sia sufficiente una buona legge delega e un buon testo unico sulla sicurezza, che sia sufficiente una maggiore cultura della sicurezza, che sia sufficiente che si cominci ad insegnare tali questioni anche nelle scuole, se non affrontiamo contemporaneamente i problemi della sicurezza sul lavoro e i temi della sicurezza del lavoro, non la garanzia della tutela della sicurezza, dell'indennità psicofisica dei lavoratori, della garanzia della tutela della loro vita. Quindi, auspico in parallelo

anche valutando il fatto che il lavoro in Commissione, e per qualche aspetto anche quello in Aula, consente di licenziare un testo che migliora il disegno di legge originario del Governo. Sono stati, infatti, ridotti i termini entro i quali il Governo dovrà esercitare la delega; è stato reso più cogente il coordinamento tra strutture sanitarie, l'INAIL e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e quindi tra prevenzione, controllo e persecuzione

l'attività delle strutture che fanno capo alla sanità e quindi alle Regioni e di altre invece, come gli Ispettorati del lavoro e l'INAIL che dipendono dai poteri dello Stato; sono state, infine, reperite le risorse per rendere possibile l'assunzione di 300 nuovi ispettori, per rendere più efficace l'azione di controllo e prevenzione, anche se - come la discussione in Aula ha dimostrato - stiamo legiferando in presenza di risorse finanziare che restano limitate. Tutto questo lavoro positivo, pur tra le difficoltà e i limiti che si sono appalesati nella discussione in Aula, a nostro parere è stato possibile anche per il lavoro svolto della Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Tofani, che ha dato con la sua attività gli elementi necessari alla Commissione lavoro per arrivare ad un risultato soddisfacente. L'impostazione generale del nostro lavoro ha contenuto entro limiti che non valicano la funzione di sussidiarietà anche il ruolo che i rapporti bilaterali tra le parti debbono avere in materia di sicurezza sul lavoro. In questo caso, infatti, quando si tratta della salute e della vita stessa delle persone, non c'è nient'altro che la norma stabilita per legge che possa esprimere una effettiva tutela. In verità, a tal proposito è emersa la maggiore ragione di contrasto, anche nella discussione in Aula e nell'intervento sugli emendamenti. Infatti, quando si tratta di sicurezza sul lavoro, le relazioni negoziali e il sistema dell'avviso comune non possono sostituire la certezza della norma, né la sua applicazione può essere modulata sulla dimensione delle imprese. La rigorosa attuazione delle misure di sicurezza sui posti di lavoro attiene infatti a quei diritti inalienabili degli individui che lavorano e che non possono essere per loro natura negoziabili e affidati ai rapporti tra le parti.

primo risultato legislativo, avvenuto sulla base di tante sollecitazioni, a cominciare da quella del Capo dello Stato, come l'avvio di un'iniziativa parlamentare sui temi del lavoro, che pongono i diritti individuali delle persone che lavorano come elementi fondativi di una nuova stagione del diritto del lavoro. Penso al superamento delle condizioni di precarietà, più volte qui ricordate, ma penso anche alla ripresa di una discussione sulle norme relative alla rappresentanza nei posti di lavoro e, perché no, alla questione che ha tanto appassionato gli anni della passata legislatura, che riguardano l'estensione dei diritti previsti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Auspichiamo pertanto una nuova stagione che punti alla valorizzazione del lavoro come condizione per la civilizzazione generale del Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il gran numero delle cosiddette che affligge il nostro Paese rappresenta una vera e propria piaga di fronte alla quale non è più possibile limitarsi alla denuncia, anche quando questa assume le forme più commosse ed indignate. Per contrastare adeguatamente il fenomeno occorre prendere decisioni, occorre reagire con forza. Ma la forza che si richiede ad una classe politica che sia realmente consapevole del suo ruolo e veramente rappresentativa del proprio Paese si può, si deve anche manifestare attraverso un cambio di passo che, con obiettività, possa partire dall'analisi di ciò che non ha funzionato per arrivare a un'impostazione originale delle soluzioni che dovrebbero essere adottate. Sono anni che si pensa di risolvere il problema degli infortuni sul lavoro con leggi che hanno una matrice formalistica ed un'impostazione repressiva. Sin dall'emanazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 gli interventi legislativi, tanto quelli che possiamo trovare disseminati un po' ovunque nella impressionante opera normativa che si è succeduta in questo periodo a qualsiasi titolo (ma che pure hanno avuto il suo riflesso sulla materia in oggetto), tanto quelli emanati *ad hoc* per recepire le direttive europee, non hanno fatto altro che continuare su questa linea, la quale, alla prova dei fatti, risulta del tutto insoddisfacente. Sono aumentati gli adempimenti burocratici e sono state inasprite le sanzioni, eppure il tragico fenomeno di cui siamo qui a parlare non ha ancora invertito il proprio *trend*. Cosa dobbiamo fare se nonostante queste leggi il numero degli infortuni e delle morti rimane sostanzialmente costante? Occorre che la classe politica sappia assumersi la responsabilità di abbandonare schemi mentali e derive ideologiche del tutto anacronistiche per aderire a impostazioni e prospettive che siano maggiormente aderenti alla realtà lavorativa del nostro Paese, alle condizioni di salute e sicurezza in cui questa si svolge. Non si tratta tanto di biasimare il passato. L'occasione è di quelle che non meritano la solita avvilente strumentalizzazione e le solite polemiche sterili tra maggioranza e minoranza. Si tratta soprattutto di interpretare la necessità di rinnovarsi e di proporsi come promotori di risposte concrete alle esigenze reali di un Paese che abbiamo l'onore di rappresentare. Se ciò significa per ciascuno di noi fare i conti con il proprio retaggio culturale, e quindi anche politico e legislativo, difficilmente oggi potremmo trovare occasione più nobile e dignitosa. In tal senso, mi permetto di citare le parole che un nostro collega, il senatore Tofani, ha pronunciato in apertura del dibattito in quest'Aula: «Bisogna comprendersi, bisogna osare». Una felice espressione che illuminava lo spirito di quello che avrebbe dovuto essere un dibattito sereno nei confronti di un impegno pressante e non più eludibile. Ciò nonostante ci troviamo oggi ad esprimere un voto sul disegno di legge che concede una delega al Governo per il riassetto dell'intera materia in esame il cui contenuto, a fatica, può essere definito veramente innovativo. Sebbene in Commissione si sia dato luogo ad un dibattito sereno, non si può dire che il lavoro in Aula abbia fornito le risposte attese, anzi sembra che il disegno di legge abbia seguito una deriva involutiva: troppi vizi continuano ancora a svalutare il risultato normativo che andiamo a votare. Innanzi tutto, non condividiamo l'impostazione generale di un testo che da un lato impone tutta una serie di norme immediatamente vincolanti e, dall'altro, conferisce al Governo una delega, invero troppo generica, per il riassetto e la riforma della normativa vigente. Ci sarebbe da discutere sulla forza cogente delle norme previste in questo disegno di legge. Ci chiediamo quanto imbarazzo potrebbe provocare nella maggioranza l'esercizio della delega da parte del Governo che possa andare eventualmente nel senso contrario, magari di soppressione, di tali norme. Ma non è questo il punto. Ci saremmo aspettati ben altra soluzione, ovvero la realizzazione di un sistema organico della prevenzione piuttosto che un semplice testo unico, quasi una raccolta legislativa che si limiti ad armonizzare e solo talvolta a semplificare, mai comunque a ridurre, le più varie disposizioni. Avremmo voluto discutere dei criteri specifici per realizzare l'architettura complessa, ma razionale, di un impianto normativo rinnovato nel suo spirito più profondo, dove gli organi istituzionali possano operare in modo integrato, dove gli istituti nazionali possano collaborare secondo le proprie specifiche funzioni, ma soprattutto dove le imprese, i lavoratori e tutti i soggetti coinvolti nel sistema produttivo non siano più ridotti ad oggetto passivo di norme, sanzionatorie o risarcitorie, ma possano aspirare ad un pieno coinvolgimento come soggetti attivi, finalmente promotori della cultura della prevenzione. Di tutto questo nel disegno di legge non se ne vede traccia, ma anzi è possibile scorgere un avvitamento sui consueti, verrebbe da dire antichi, difetti che hanno afflitto la normativa vigente e sui quali torneremo successivamente; perché, prima ancora della loro analisi critica, ci preme sottolineare quello che noi consideriamo il vero punto dolente di questo testo, ovvero il termine per l'esercizio della delega. Non è possibile sottacere la lentezza del processo posto in essere né sminuire la sua drammatica portata. Si doveva procedere senza indugio verso una quanto più rapida definizione dell'intera materia ed invece si è assistito ad uno sconcertante balletto di termini. Con il termine di nove mesi, di cui al primo comma dell'articolo 1, nella migliore delle ipotesi, considerando anche il susseguirsi dei futuri passaggi in Aula, ma soprattutto tacendo di tutte le possibili insidie, non riusciremo ad avere un testo definitivo prima della metà del prossimo anno. Un ritardo assurdo e irresponsabile del quale, pur con tutta la buona volontà, non siamo riusciti a capire le ragioni, a meno che queste non vadano cercate nella misera esigenza di trovare i fondi per sostenere tutte le prevedibili voci di spesa. Una ricerca affannosa, che il Governo forse non aveva preventivato e che oggi deve porlo in serio imbarazzo, tanto da posticipare oltre il limite della decenza l'esercizio della delega. Il riferimento al profilo soggettivo della materia ci permette di introdurre quello che a nostro avviso è uno dei grandi assenti del disegno di legge, ovvero la micro, la piccola e la media impresa. Mi chiedo ancora una volta come sia possibile pensare di rinnovare l'approccio alla salute e alla sicurezza del lavoro in Italia senza cogliere in tutte le sue implicazioni le specificità di tali soggetti. Di fronte a eguali rischi e pericoli, infatti, la loro capacità di prevenzione e di risposta rimane drammaticamente diversa e non può essere altrimenti. L'estensione indiscriminata delle norme a tutti i soggetti quale che sia la loro dimensione aziendale rappresenta un'imposizione insostenibile per i destinatari, la cui efficacia peraltro nei confronti dei lavoratori è assai dubbia. Non credo che le massime autorità del nostro Paese - a partire dal Presidente della Repubblica o dallo stesso Presidente del Senato, che ha voluto appositamente istituire una Commissione d'inchiesta, solo per fare un esempio io non credo, dicevo, che questi volessero solo fare un mero richiamo formale alla sensibilità generale di noi parlamentari, ovvero dotarsi di uno strumento di indagine storica o statistica, quanto piuttosto chiedere con autorevolezza una risposta concreta ad una tragedia cui si deve porre fine il più velocemente possibile. Ed invece sembra che siamo qui a contare i giorni in attesa che, negli oscuri meandri della contabilità nazionale, si scopra per caso qualche residuo di cassa

che non sono state eccepite in questa sede nella speranza che l'Aula recepisse il gesto di buona volontà e che proprio per la vostra ignavia permangono sul futuro del testo come una imbarazzante spada di Damocle. se anche si volesse superare la portata negativa di tali pregiudiziali, come abbiamo comunque fatto, altri sembrano i difetti di questo disegno di legge. Ci aspettavamo di arrivare all'emanazione di un disegno di legge che potesse dare un diverso tipo di risposte, che avesse finalmente compreso il significato e l'importanza dell'informazione e della formazione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Dobbiamo invece rammaricarci dell'occasione perduta. Il testo oggi emanato sembra zoppicare dal punto di vista costituzionale.

in materia di formazione e prevenzione. Per tutti questi motivi, ci troviamo ad esprimere il voto non favorevole del nostro Gruppo e lo facciamo con l'amarezza di chi ha visto quest'Aula sprecare l'occasione di dare un segnale importante al Paese.

pone una questione che non è solo quella della sicurezza delle condizioni di lavoro, ma anche quella della qualità dell'impresa nel nostro Paese.

un processo di qualificazione e di tutela della condizione di lavoro. Sono state dette in quest'Aula molte cose che richiederebbero più tempo rispetto a quello che ho a disposizione,

che però ha ancora la necessità di maggiori risorse, che il Governo si è impegnato a mettere in campo per consentire un rafforzamento della prevenzione degli infortuni sul lavoro. a concludere, che con questo voto favorevole stiamo mettendo il Parlamento in connessione sentimentale con il Paese e le sue condizioni e ridiamo dignità al lavoro attraverso una più forte tutela delle sue condizioni di sicurezza.

perché abbiamo, in realtà, condiviso l'esigenza di una legge delega per produrre un testo unico in parte compilativo, ma in parte anche innovativo in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Già nella scorsa legislatura, peraltro, ci fu una netta contrapposizione tra l'impostazione prodotta dalla Casa delle Libertà, attraverso il proprio disegno di legge delega, contenuto nel più ampio provvedimento rivolto alla semplificazione della nostra normativa, e la posizione che la coalizione di centro-sinistra, allora di opposizione, ebbe nei confronti di quel disegno di legge e successivamente del testo unico che in relazione ad esso fu prodotto. Si contrapposero, insomma, due impostazioni, le stesse due impostazioni che si sono contrapposte nel corso dell'esame di questo provvedimento. Per la Casa delle Libertà il testo unico nasce da un'esigenza di semplificazione, di adattamento della norma soprattutto alla piccola dimensione d'impresa, posto che la disciplina vigente è stata costruita tutta sull'impresa di maggiore dimensione, sull'impresa strutturata; nasce, inoltre, da un'esigenza di coinvolgimento delle parti sociali attraverso la bilateralità, cioè quegli organismi che le parti sanno produrre ove cooperano soprattutto con riguardo a quel bene primario che è la salute e sicurezza del lavoratore; nasce, infine, dalla volontà di produrre un approccio per obiettivi mediante, ad esempio, l'impiego delle norme di buona tecnica o le buone prassi. Noi siamo, insomma, animati dal volere confrontare le norme con la realtà e con i risultati che possono ragionevolmente essere prodotti, tanto che abbiamo insistito nel volere un sistema di monitoraggio condiviso da Stato e Regioni come da imprenditori e lavoratori, in modo da costituire esso un utile strumento per l'orientamento della quotidiana azione politica e amministrativa idonee a contrastare il fenomeno delle morti, degli infortuni e delle malattie sul lavoro. Per l'Unione, in realtà, il testo unico sembra necessario solo per l'obiettivo di rafforzare i vincoli formali e le sanzioni a carico dell'impresa, indistintamente di tutta l'impresa, di tutte le imprese. Alla base di questa impostazione, infatti, che inesorabilmente l'impresa sia fisiologicamente il luogo dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ora, nel corso del confronto parlamentare il dialogo, in realtà, non c'è stato

è stata prodotta; nessuna modifica dell'apparato sanzionatorio, assolutamente destinato ad essere ineffettivo, è stata accolta; nessuna fiducia è stata espressa nei confronti della bilateralità e quindi della collaborazione

Abbiamo a malapena condiviso l'esigenza di rafforzare i controlli, posto che il Governo Berlusconi aveva riformato le funzioni ispettive e bandito il concorso per circa 900 ispettori aggiuntivi, che in parte qui fortunatamente procediamo ad assumere. In conclusione, non possiamo condividere un provvedimento che nei suoi criteri e nei suoi principi contiene ragionevolmente una maggiore pressione burocratica sulle imprese, ulteriori elementi di aleatorietà nella vita dell'impresa, una ragionevole ineffettività delle norme per contrastare infortuni e malattie, là ove più si producono, là ove più dovrebbero essere contrastati. Per tali ragioni, insisto, non possiamo condividere questo provvedimento. Signor Presidente, in cinque minuti è difficile racchiudere le speranze e le delusioni di questi mesi. di speranze e delusioni che si sono sommate da quando il provvedimento è stato assegnato al Senato. Non posso non ricordare l'impegno e l'entusiasmo profuso per fare in modo che la Commissione

e per fare in modo che un tema così importante potesse trovare il massimo della convergenza.

o comunque di grande soddisfazione e di grande condivisione. Mi auguro che nel percorso successivo alla Camera venga rivisto quanto è stato definito in questa Aula. Lo dico con rammarico, per non

Quindi, signor Presidente, colleghi senatori (concludo il mio intervento, perché credo di aver esaurito il tempo che lei cortesemente ha voluto concedermi), trionfa in me, nel Gruppo Alleanza Nazionale, in questa fase, una grande delusione, perché non è stato accolto quell'appello che, prima ricordavo, rivolto dalle più alte autorità dello Stato e non si è capito - perlomeno io non l'ho capito - perché si è voluto irrigidire questo rapporto non dando una soluzione che poteva essere condivisa.

al Paese, ai lavoratori, alle persone che lavorano ed alla robusta sollecitazione che il Presidente della Repubblica più volte ha fatto perché il Parlamento adeguasse in modo rapido la normativa di contrasto e di prevenzione al fenomeno così difficile da estirpare nella vita del nostro Paese, nella vita delle persone che lavorano in questa nostra Italia. Tre parole chiave dicono di questo provvedimento: razionalizzazione, contrasto, prevenzione. Razionalizzazione, semplificando le norme e portando a compimento un apparato normativo attraverso la delega al Governo, che dia un quadro generale di norme che siano effettivamente legate all'ambito comunitario e siano legate ai cambiamenti che sono avvenuti nelle imprese; di contrasto, che si è manifestato in particolare nell'evidenziazione dei diritti essenziali delle persone che lavorano, in particolare di quelli più deboli, le donne e gli immigrati; di contrasto attraverso una normativa diversa sugli appalti ed i subappalti, dove si verificano la gran parte degli incidenti mortali; di contrasto attraverso un aumento degli ispettori del lavoro che fanno le verifiche ed i controlli sulle imprese. La terza parola chiave è prevenzione, perché gli incidenti sono evitabili, specialmente quelli mortali. Investire sulla prevenzione attraverso tre vie: la formazione sperimentale sperimentale nel campo della formazione professionale, la formazione nelle scuole con un cinque per cento di tempo dedicato alle materie giuridiche e tecniche, il credito di imposta per quelle imprese che investono in percorsi formativi certificati per i lavoratori. Un significativo investimento di risorse: 20 milioni di euro in più per assumere 300 ispettori che si aggiungono ai 300 già assunti con la finanziaria, la più massiccia manovra di inserimento di nuove persone che facciano controlli e contrasto nelle imprese; 20 milioni nuovi di credito di imposta per quelle imprese che fanno formazione per i lavoratori e 20 milioni per le scuole, per la formazione professionale in forma sperimentale. Sono 60 milioni di risorse che vengono destinate al contrasto, alla prevenzione, alla razionalizzazione delle norme. credo che questo lavoro dia il significato di un testo che appare armonico e capace di darci una normativa solida nel campo della sicurezza del lavoro. Il rispetto della vita e della dignità delle persone passa anche da questo provvedimento. L'Ulivo esprime convintamente il suo voto favorevole.

il comma 17-*bis* dell'articolo 3 stabilisce che entro il 30 giugno 2007 il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni internazionali, che sono state rinnovate con vari provvedimenti e con la legge che converte il citato decreto-legge. a tutt'oggi nulla risulta, né alla Commissione esteri né alla Commissione difesa, quanto meno in questo ramo del Parlamento. Credo che questo sia un fatto veramente grave, perché sulla principale e più delicata attività che svolge il nostro Paese all'estero il Governo è inadempiente rispetto a una disposizione di legge alla quale bisognerebbe adempiere in ogni caso. Non è neppure necessario, ma ritengo sia doveroso, ricordare che in questi giorni la situazione, in

non venir meno a quanto la legge impone. La scadenza era il 30 giugno e purtroppo mi sembra inverosimile rispettarle. Pertanto, le chiedo di sollecitare il Governo ad adempiere a una disposizione di legge, specialmente in questo momento delicato.

vorrei richiedere una risposta urgente. L'interpellanza ha come tema e argomento principale la Conferenza internazionale sulla giustizia, che si svolgerà il prossimo 3 luglio a Roma. A maggior ragione c'è una richiesta di risposta urgente, essendo stata